Restano peraltro accantonati gli emendamenti agli articoli 7, 30, 32, nonché gli aggiuntivi agli articoli 8 e 12 riportati nel fascicolo 4. Colleghi, o si prende posto e si cessa questo brusìo e questa disattenzione quando si deve riferire sui pareri delle Commissioni oppure, se vogliamo procedere su un tema così importante a successivi rinvii e a successive sospensioni della seduta, basta mettersi d'accordo.

ribadisce il parere espresso in data 14 gennaio 2009. Ritiene pertanto necessaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

ai sensi della medesima norma costituzionale - e dell'emendamento 55.500 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo di copertura». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di proprio competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 35.0.800/2, 35.0.800/6, 35.0.800/7 e 35.0.800/8. In ordine alla proposta 35.0.800 il parere è non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano inserite, in fine, la parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio". Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative».

Signor Presidente, in una scorsa seduta avevo sollevato dei problemi di copertura in relazione al fatto che l'articolo 19, così come votato dall'Assemblea, che aveva sostituito l'originario articolo 9 del disegno di legge, introduce un duplice profilo di reato: il reato di ingresso illegale e il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato. la copertura finanziaria finanziaria per la modifica delle ipotesi di reità, che aveva aumentato la platea dei destinatari dei processi penali, non poteva più essere quella riguardante l'originario articolo 9 - che introduceva esclusivamente il reato di ingresso illegale - e doveva essere

da qui a quando arriveremo all'articolo 55 c'è il tempo e la necessità di compiere questo approfondimento, fermo restando che il suo intervento specifico potrà farlo su questo aspetto. LI GOTTI *(IdV)*. Quindi devo sviluppare le osservazioni o no?

lei, correttamente, per ragioni legate all'economia del nostro lavoro, ha rinviato l'esame di questo tema all'articolo 55. Tuttavia, siamo in presenza di un rilievo, quello del senatore Li Gotti, già formulato diffusamente in una precedente seduta che ha già avuto un suo *iter*. Il Presidente del Senato, infatti, allorquando il senatore Li Gotti sollevò un serio problema di copertura relativamente all'articolo 19, ebbe ad accantonare tale articolo, rinviando la questione in Commissione bilancio e sollecitando un riesame dei profili di copertura. La Commissione bilancio in data di ieri ha esaminato nuovamente a maggioranza ha ritenuto di dover confermare il parere favorevole. I Gruppi di opposizione in quella sede hanno formulato pesanti rilievi su questo punto; io adesso non voglio affrontare il merito,

e fondato rilievo. Parliamo infatti di profili di copertura, legati all'introduzione di questa nuova fattispecie di reato, che si basano su un dato fornito dalla Ragioneria generale dello Stato palesemente falso.

chiaramente sottostimato, si pone un problema serio e quindi, nell'accogliere la sua decisione, signor Presidente, le proporrei però di integrarla, nel senso di invitare il Governo

rispondendo al senatore Li Gotti, era proprio questo. Il presidente Schifani aveva già rinviato tale aspetto alla Commissione e proprio questa mattina è stato letto il parere della Commissione, a cui lei faceva riferimento,

per non ostacolare i lavori nel momento in cui si riprenderà con l'esame degli emendamenti accantonati, vorrei depositare la proposta di riformulazione per dare il tempo alla

parere del Governo

di inserire, dopo la frase: «La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati», la seguente: «, il quale decide entro dieci giorni».

Presidente, nella seduta in cui abbiamo trattato il tema dei testimoni di giustizia abbiamo affrontato un argomento molto delicato

l'inserimento, ad alcune condizioni, nella pubblica amministrazione. È stato sollevato dal Governo il problema serio della sicurezza; è un tema che non deve essere trascurato

di fare una ulteriore correzione al testo che prevedeva l'assunzione nella pubblica amministrazione, così come formulato da parte del Partito Democratico. Abbiamo pensato che quella legittima preoccupazione sulla sicurezza potesse essere recepita, prevedendo la possibilità - e non quindi un diritto soggettivo - di un inserimento, tenuto conto del cambio di generalità che può soddisfare le esigenze di riservatezza e di protezione del testimone, nella pubblica amministrazione, presso il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici, dove è possibile organizzare con un decreto apposito il tema della sicurezza e garantire quindi questo aspetto. È una preoccupazione comune e condivisa. Ecco perché invitiamo il Governo ad accettare questa riformulazione in modo da poter così condividere un percorso tanto atteso, che ci mette nelle condizioni di risolvere casi che stanno diventando molto preoccupanti e, nello stesso tempo, di non violare quel principio di sicurezza a cui il Governo si rifà.

dei subemendamenti ad esso riferiti. Vorrei segnalare all'Aula, affinché rimanga agli atti, che si tratta di una materia molto delicata concernente l'attività di organizzazioni, associazioni o movimenti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

della quale veniva ripercorsa la struttura. Ricordo che la legge Mancino, in particolare all'articolo 3, prevedeva che dopo una sentenza irrevocabile di accertamento della natura terroristica o eversiva dell'associazione potesse intervenire un provvedimento del Ministro dell'interno per stabilirne lo scioglimento. La legge Mancino prevedeva su questa linea che nei casi particolarmente gravi, in via cautelativa,

o l'opportunità di sciogliere queste organizzazioni eversive; allo scopo sarebbe dovuto intervenire il giudice competente entro dieci giorni ed entro dieci giorni sarebbe stato possibile presentare ricorso in Cassazione. L'impostazione originaria dell'emendamento 33.0.600 invertiva in questo secondo caso l'ordine degli interventi, nel senso che sarebbe stata la magistratura a segnalare al Ministro, anche in via cautelare e preventiva, quindi doveva essere un provvedimento del Ministro a decidere della questione. Questa pausa è stata sicuramente utile per una riflessione da parte di tutti noi, sia nelle Commissioni che anche con il Governo, per fare in modo che venga riprodotta tale e quale in questo testo e nei subemendamenti la struttura della legge Mancino, a favore della quale, ricordo, nel 1993 votò, quasi all'unanimità,

In questa disciplina si stabiliva che la sospensione

si stabiliva che il provvedimento dell'autorità giudiziaria, cioè del tribunale competente per i reati per cui si procedeva, fosse sottoposto a

si toglie potere alla magistratura per darlo al Ministero, tenendo presente che comunque, quando c'è una sentenza passata in giudicato, già prima si prevedeva che fosse il Ministero a stabilire lo scioglimento definitivo dell'associazione.

avvertita. Tradizionalmente i fenomeni criminali riferibili al crimine organizzato e quelli riferibili al terrorismo sono

a metodi tipici della criminalità organizzata e alcune indagini hanno portato proprio in questa direzione: basti pensare all'indagine sulla 'ndrangheta e sui rapporti che essa aveva con i cartelli colombiani

che nell'ampia accezione di crimine organizzato si intendano sia la criminalità organizzata tipica sia il terrorismo. Vi sono diversi provvedimenti delle autorità europee

hanno dato vita ad un modello europeo che comprende in modo indistinto i fenomeni criminali di terrorismo e quelli riferibili alla criminalità organizzata.

avere un organo centralizzato per la criminalità organizzata rappresentato dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Procura nazionale antimafia, cosa che invece non esiste per i reati di terrorismo. Ciò crea grandi problemi.

viene segnalata la difficoltà di indagine e di rapporto con gli altri Paesi europei quando si tratta di fenomeni così strettamente connessi.

di criminalità organizzata, affidato al medesimo organo che già cura questi affari, anche se in modo estremamente complesso. Basti pensare che nel momento in cui ci si rapporta con l'Europa per i problemi di terrorismo non esiste un unico interlocutore italiano, ma esistono 26 procure distrettuali.

Poche settimane fa, nel 2008, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura è venuto in Italia per accertare le condizioni di detenzione dei reclusi sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis*. La modifica che ci è stata proposta dalle Commissioni vuole allungare il regime duro sino a quattro anni, prorogabili all'infinito; riaprire carceri quali l'Asinara e Pianosa, chiuse tra l'altro per gli enormi costi di gestione; invertire l'onere della prova della pericolosità, facendola gravare sul detenuto. Essa inoltre riduce il diritto alla difesa: vengono infatti contingentati i colloqui con i difensori, dando la competenza sui reclami al solo tribunale di sorveglianza di Roma, violando con ciò palesemente il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. un giudice americano della California, Sitgraves, era intervenuto per dire che in Italia vi è un rischio di tortura a causa del tanto venerato del 41-*bis* è un regime penitenziario pesantissimo e proprio a causa della sua estrema durezza la Corte costituzionale ha affermato che esso deve essere necessariamente temporaneo. L'isolamento prolungato cui i detenuti sono sottoposti produce infatti effetti irreversibili di desocializzazione e delocalizzazione; i vetri divisori ai colloqui, la negazione di ogni forma di socialità, la chiusura di ogni rapporto con l'esterno, sono giuridicamente e costituzionalmente tollerabili solo se limitati nel tempo. Eppure, purtroppo, tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra ci si indigna quando dopo 16 anni di regime un detenuto viene derubricato - questa è la terminologia carceraria utilizzata - a detenuto "Alta sicurezza" (AS): un regime poco meno duro del 41-*bis*. Pare quindi che il 41-*bis* sia l'unica arma del diritto a disposizione delle forze investigative contro la mafia. Agli inizi degli anni Novanta, cioè a pochi anni dalla sua introduzione, un funzionario dell'amministrazione penitenziaria italiana nel rispondere agli ispettori del Comitato europeo per la prevenzione della tortura di Strasburgo affermava che il regime del 41-*bis* serviva a far parlare i detenuti; una pratica che assomigliava, disse, alla tortura, una tortura che però in Italia non è reato.

di alcuni politici italiani che si sono recati in carcere non già per dare solidarietà a chi ha commesso un crimine, ma per far emergere la realtà delle nostre carceri italiane,

scritto dall'ex deputato della Rosa nel Pugno Sergio D'Elia e dall'attuale deputato radicale nella delegazione del Partito Democratico alla Camera Maurizio Turco, intitolato «Tortura democratica» e sottotitolato «Inchiesta su "la comunità del 41bis reale"». La prefazione che nella scorsa legislatura non ha potuto essere proclamato senatore, mentre sono convinto che sicuramente avrebbe recuperato molti degli argomenti che include nella prefazione a questo libro, pubblicato nel 2002. «(...) Le dure condizioni di detenzione rispondono solo ad una logica di rivalsa e a un primordiale senso di vindice giustizia. Si è risposto con Pianosa e l'Asinara alle stragi di Capaci e via D'Amelio. Il dolore dei parenti delle vittime contro le vessazioni nei confronti dei detenuti. Questo è stato messo a confronto! È giunto il momento» - ed eravamo nel 2002 - «di chiedersi che cosa è avvenuto in questi ultimi dieci anni e cosa continua ad accadere. A questo punto, non si tratta di chiedersi se le norme vigenti siano state rispettate o no, se le procedure siano più o meno corrette; si tratta di chiedersi che cosa Antimafia e Mafia stiano mutualmente facendosi fra di loro e, attraverso quella che è definita una guerra, a noi tutti. È incredibile che nessuno si preoccupi che nei confronti di, ormai vecchi, "mafiosi" i magistrati continuino a usare l'arma della tortura, dell'infamia che colpisce non solo i "mafiosi" ma sta ma sta schiacciando tutto e tutti verso la demagogia e il conformismo politico e sociale. Nessuno che consideri la gravità del fatto che i magistrati, spesso per propria impostazione ma anche per investitura pubblica e politica, più che reati di mafia, stiano perseguendo la Mafia-istituzione, sicché invece di investigare reati specifici, produrre prove e fare i processi, stiano in realtà producendo (assieme alla mafia, com'era naturale prevedere) pentiti e offrendo esempi alla pubblica riprovazione. Il conformismo dell'Antimafia, quella parlamentare e quella della cosiddetta "società civile", sta facendo strame di stato e di diritto, di legalità e di umanità, di società e di persone. Eppure, il 41 bis non si discute. Chi ne tocca i fili, le corde cui si impiccano detenuti così come la legalità, muore? Questa estate,» - nell'estate del 2002, appunto «nei giorni della loro "protesta pacifica e civile",» - e forse alcuni di voi ricorderanno cosa avvenne quell'anno all'interno di molte carceri italiane - «i detenuti in 41 bis si sono rivolti alle più alte cariche dello Stato, in questi termini:» e qui cito un documento che fu fatto circolare allora: «"Stiamo mettendo in atto un Satyagraha che non mira certo alla abolizione del regime del "carcere duro" (compito questo, in una società democratica, di esclusiva competenza del Legislatore), bensì al rispetto delle regole, delle norme vigenti, nonché al rispetto della dignità umana che quotidianamente viene calpestata e umiliata". Loro, i fuorilegge, hanno manifestato nelle carceri per il rispetto della legalità; nel frattempo, nessun tutore della legge si è manifestato contro fuorvianti applicazioni, nessun legislatore si è levato in Parlamento per dire che il "41 bis reale" è una barbarie e che questa - non chissà quale altra - si vuole eternizzare.

lotta non violenta, condotta con uno sciopero della sete di 7 giorni di Pannella e uno sciopero della fame di centinaia di detenuti che, con le parole che ho appena citato, lo sostenevano, si arrivò ad una decisione adottata dalla Camera dei deputati in cui si prese atto dell'impossibilità di ratificare l'elezione di 12 parlamentari della Repubblica. Concludo l'illustrazione del perché riteniamo che non si debba insistere non soltanto con il 41-*bis*, ma sicuramente nel proporre come misura di lotta alla mafia l'indurimento di un qualcosa che negli ultimi anni non ha dato i risultati sperati, con quest'ultima citazione, sempre dalla menzionata prefazione al libro: «L'opera, l'inchiesta, la fatica e la tenacia di Maurizio Turco e di Sergio D'Elia» - che all'epoca non erano parlamentari - «costituiscono un evento, approdo e sintesi di uno dei percorsi radicali nelle caienne delle istituzioni e della società italiana. Ora ciascuno» questo libro può essere scaricato dal sito nessunotocchicaino.it, perché non è più stato ristampato ristampato «potrà meglio intendere la continuità, l'intimità profonda e attualissima della "comunità *reale* del 41 bis *reale"* con i luoghi, che si ritenevano e ritengono scomparsi, delle "deportazioni" di veri o presunti criminali, condannati alla "morte (per intanto) civile"».

Non siamo pregiudizialmente contrari al testo licenziato dalle Commissioni. Il testo che abbiamo ritenuto di proporre con il nostro emendamento ricalca alla lettera quello elaborato dagli uffici della Procura nazionale antimafia così come ci è stato consegnato in Commissione giustizia, in cui vengono affrontati i punti critici dell'attuale sistema. Il testo che ci è stato affidato per la valutazione dalla Procura nazionale è stato certamente preso in considerazione prima dalla Commissione giustizia e poi dalle Commissioni

due osservazioni critiche. È certo che il nostro Paese non può non dotarsi di

anche se sappiamo perfettamente, per le conoscenze che nel corso degli anni si sono accumulate, che esiste una mafia dietro le sbarre

vuole avere maggiore agibilità e non essere subalterna ai mafiosi in carcere. è sempre stata questa insofferenza della mafia libera che gradisce una maggiore durezza nei confronti dei mafiosi in carcere. Il testo licenziato dalle Commissioni è sicuramente nella direzione di una maggiore durezza: ben venga; però il rischio che corriamo è che quando si vuole essere troppo duri si commettano poi degli errori. L'articolo 25 della Costituzione fissa un principio insuperabile qual è quello del giudice naturale. L'ordinamento penitenziario, che prevede l'articolo 41-*bis*, individua anche il giudice competente a decidere sui provvedimenti applicativi e sulle proroghe. Il giudice competente è individuato nel tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto internato è assegnato. Questo nel rispetto dell'articolo 25 della Costituzione. Nel testo proposto, che noi vorremo sostituire con il nostro emendamento, si dice invece che la competenza per decidere sul particolare regime e, quindi, sui reclami avverso i provvedimenti applicativi

Roma. È vero che per altre fattispecie vi è una norma analoga. Per esempio, per i collaboratori di giustizia in materia di benefici penitenziari

determinata dalla pericolosità della rilevazione del luogo di detenzione e dal fatto che i collaboratori di giustizia per legge hanno il loro domicilio in Roma. Questo prevede la normativa sui collaboratori di giustizia. Estendere, invece, anche per l'applicazione e per il reclamo avverso il regime del 41-*bis*, ad un unico giudice derogando al principio costituzionale dell'articolo 25 espone la norma così proposta a profili di radicale incostituzionalità. Noi dobbiamo essere attenti: essere duri e rigorosi è una cosa, essere rispettosi del nostro ordinamento è un'altra, perché essere troppo duri significa inserire un *vulnus* nell'articolo 41-*bis* che potrebbe essere dichiarato incostituzionale per violazione dell'articolo 25 della Costituzione. Io richiamo alla delicatezza di questo passaggio. Facciamo le norme dure, ma evitiamo che le stesse possano incorrere in una violazione di un precetto costituzionale perché, diversamente, dall'esistenza di una norma ci troveremmo con un vuoto normativo. Ecco perché abbiamo sollecitato quel nostro testo, pur apprezzando il testo licenziato dalle Commissioni, se non per la parte che assegna ad un unico giudice, ossia a quello di Roma, tutta la competenza per i reclami provenienti da qualsiasi parte d'Italia. Sollecito, quindi, una riflessione del Governo e dei proponenti di quel testo perché riteniamo valide le intenzioni, ma pericolosi gli effetti

il signor Presidente dovesse cogliere segnali in questo senso, per la possibilità di arrivare ad un testo condiviso che rimedi ai rischi di incostituzionalità. *(Applausi Signor Presidente, anche noi abbiamo proposto un'ipotesi di sostituzione del testo dell'attuale articolo 41-*bis*, che ovviamente è in sintonia con quanto detto in precedenza dal collega Li Gotti e che tiene conto del confronto che si è avuto in Commissione

gli effetti negativi che sono stati monitorati in questi anni e che sono legati a quella giusta decisione che il Parlamento assunse di stabilizzare il regime carcerario del 41-*bis*. da affrontare oggi è come sia possibile, e in che termini sia possibile, rendere più efficace questo regime carcerario. Infatti, è efficace se e in quanto elimina ogni forma di collegamento tra il detenuto mafioso e le organizzazioni e le organizzazioni criminali sul territorio: se non produce questo effetto determina un'inutile compressione dei diritti di libertà e, quindi, espone ad un rischio di incostituzionalità superiore una norma che oggettivamente prevede un regime di sicurezza molto stretto. Pertanto, noi dobbiamo farci carico dell'esigenza di contemperare l'interesse generale a che questo regime restrittivo sia funzionale a estirpare ogni tipo di collegamento, di di *leadership* interna alle carceri nei confronti delle organizzazioni criminali. Allo stesso modo, dobbiamo verificare come ciò in concreto sia avvenuto in questi anni e quali possono essere i correttivi. Tra questi ne abbiamo segnalato alcuni, faccio qualche esempio perché non voglio ripetere cose già dette che condivido: anzitutto rafforzare il ruolo della Procura nazionale antimafia, perché è chiaro che non è sufficiente il compito di coordinamento e di conoscenza che la Procura ha nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata. Si avverte la necessità di un intervento più efficace e penetrante anche nel potere di iniziativa, di proposta e di verifica del regime carcerario, così come la necessità di intervenire nella fase che riguarda l'interpretazione delle disposizioni. Vi è infatti un contrasto tra l'orientamento della Corte di cassazione su questa materia e l'orientamento che, viceversa, hanno diversi tribunali di sorveglianza, con la inevitabile

di intervenire anche sul sistema di controllo del detenuto e sulla valutazione del pericolo del collegamento. Il riferimento che viene fatto alla Il riferimento che viene fatto alla cosiddetta capacità di mantenere i contatti ha prodotto dei risultati anche sotto il profilo di alcune decisioni dei tribunali di sorveglianza, che sono in controtendenza rispetto allo spirito della norma. La necessità che si pone, viceversa, è quella di verificare costantemente se sussista in concreto il pericolo di possibili collegamenti tra il detenuto e le associazioni criminali. Queste sono alcune delle ragioni che ci portano, pur apprezzando lo sforzo che è stato fatto in Commissione per migliorare il testo, a chiedere anche noi un voto favorevole ai nostri emendamenti, che vanno nella direzione di fornire agli organi preposti alla prevenzione, al contrasto e al controllo maggiori strumenti e di rendere più effettiva, a fronte di una grande compressione dei diritti di libertà che impone il regime carcerario del 41-*bis*, la

Presidente, affrontiamo adesso con il 41-*bis* un punto prezioso e delicato della lotta alle mafie. Il 41-*bis* - i colleghi lo sanno - è stata una grande intuizione di Giovanni Falcone, una grande intuizione su cui non penso possa valere quella infausta distinzione che in altri anni abbiamo utilizzato nella lotta al terrorismo, cioè il principio dell'equidistanza, mafia - in questo caso - e antimafia, perché in un Paese democratico non può esserci un'impostazione equidistante. Il Partito Democratico sta con tutte le formazioni politiche democratiche nell'antimafia e il 41-*bis* è una grande risorsa della nostra democrazia, così come lo pensò Falcone e come poi è stato attuato. E' una grande risorsa della nostra democrazia perché le organizzazioni mafiose sono le uniche organizzazioni criminali in grado di esercitare il loro dominio, le loro attività, anche le più terribili, drammatiche e violente, anche quando i loro boss si trovano all'interno del sistema carcerario. Lo intuì Falcone: i boss mafiosi considerano il carcere una porzione del loro territorio da controllare, su cui esercitare il loro dominio

sono sempre riusciti, dal carcere, a non sospendere mai la loro attività criminale, a stabilire chi bisogna uccidere, a partecipare alle scelte sulle stragi a stabilire quale operatore economico estorcere, quale appalto o subappalto truccare e - perché no - quale politico votare.

che le organizzazioni mafiose non mettono in sospensione il capo, il boss, quando viene catturato. Egli rimane in testa a quell'organizzazione (alla famiglia se è Cosa nostra, alla 'ndrina o alla famiglia camorrista)

la funzione di vertice dell'organizzazione mafiosa. Falcone intuì queste due dimensioni: le organizzazioni mafiose considerano il carcere una porzione del loro territorio su cui imporre il loro dominio dal carcere, continuano ad esercitare la loro violenta e drammatica funzione di comando verso l'esterno. Ecco perché

Ecco perché, colleghi, vi è bisogno di intervenire e di rendere più rigoroso il 41-*bis*. Le proposte che abbiano avanzato vanno in questa direzione e la sintesi che è stata trovata in Commissione va in tale direzione. Abbiamo proposto un periodo di tempo più lungo proprio perché l'appartenenza è totale e l'organizzazione non sospende mai la propria attività. Abbiamo proposto anche di utilizzare delle particolari carceri che non sono speciali. Pensate un po', colleghi: nelle isole minori ci sono delle carceri per detenuti comuni.

nella proposta si avanza l'ipotesi di riaprire Pianosa e l'Asinara dove i costi sono inferiori e dove la funzione rieducativa prevista dalla nostra Costituzione può diventare realtà, dove naturalmente è più semplice per lo Stato impedire la comunicazione devastante verso l'esterno. Vi è un punto, cari colleghi, accanto all'insieme di norme

prevedevamo un'altra soluzione, quella del giudice della misura di prevenzione personale nel distretto in cui è stato giudicato il *boss* mafioso, perché coerente con l'impostazione che abbiamo dato della misura di prevenzione, coerente con l'inversione dell'onere della prova, con la conoscenza che quel giudice ha Il Governo ha fatto un'altra scelta: ha pensato di indicare il giudice di sorveglianza del tribunale di Roma.

anche di efficacia di gestione del 41-*bis*. Abbiamo invitato il Governo in questi giorni a rivedere questo aspetto; il Governo lo ha mantenuto. Comunque,

che sono il frutto della nostra proposta e di quelle che i relatori hanno avanzato in Commissione e che ci mettono in condizione di avere finalmente, intorno al 41-*bis*, una soluzione efficace e seria, duratura, in grado di superare quel limite che abbiamo riscontrato in questi anni nell'attuazione del 41-*bis*. Colleghi, è un momento questo molto importante. Bisogna avere il coraggio di colpire al cuore le organizzazioni mafiose, di non limitarsi a contenere la loro portata criminale, ma di provare a dotarci nella nostra democrazia, con le regole e le garanzie previste nella Costituzione e nelle norme della nostra democrazia, ad eliminare le organizzazioni mafiose

con sentenze passate in giudicato. Semmai, cari colleghi, ci dovremmo interrogare sulla durata delle pene, che oggi sono estremamente al di sotto della portata della minaccia delle organizzazioni mafiose. Avanzeremo a tal proposito delle proposte in modo tale da evitare quello che tutte le indagini di mafia ci dicono, cioè che dopo pochi anni

Ecco perché su questo punto ci siamo: dobbiamo apprezzare la scelta che in Commissione è stata compiuta, la convergenza che è stata realizzata. Ne siamo fieri, perché siamo in sintonia, tranne per quanto riguarda la misura

per eliminare le mafie, per cancellarle ed evitare che possano continuare a costituire una minaccia per la società, la democrazia e molti territori del nostro Paese.

intende introdurre un articolo aggiuntivo che prevede un nuovo reato nel nostro codice penale. Può sembrare singolare il fatto che dei radicali propongano un nuovo reato, ma

Intendo ora leggere una citazione di Antonio Cassese, contenuta nelle sue memorie di presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti. È una dichiarazione

«È stato facile stabilire un primo punto fermo, cosa debba intendersi per tortura. Su questo punto ci soccorrevano la storia, gli scritti dei grandi illuministi (Verri, Beccaria, Voltaire, Manzoni), le letture recenti (ad esempio, "La *Question*" di Henri Alleg, sulla guerra di Algeria o "La Confessione" di Artur London, in cui il dirigente politico cecoslovacco descrive gli orribili metodi con cui i servizi di sicurezza del suo Paese torturavano i dissidenti politici negli anni Cinquanta); ci sono state di grande aiuto anche le sentenze della Corte europea sui diritti dell'uomo (ad esempio quelle sulle cosiddetti tecniche di aiuto all'interrogatorio, usate dagli inglesi nell'Irlanda del Nord) o il rapporto della Commissione europea sui diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli. Senza nemmeno discuterne tra noi, ci è sembrato evidente che la tortura fosse qualunque violenza o coercizione, fisica o psichica, esercitata su una persona per estorcerle una confessione o informazioni, o per umiliarla, punirla o intimidirla. Nella tortura la disumanità è deliberata: una persona compie volontariamente contro un'altra atti che non solo feriscono questa ultima nel corpo o nell'anima, ma ne offendono la dignità umana. Nella tortura c'è insomma l'intenzione di umiliare, offendere

Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, del 1984, ha definito chiaramente cosa si debba intendere per tortura,

informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o sottoporla a coercizione, per qualunque ragione basata su una discriminazione di qualsiasi tipo, a condizione che il dolore o la sofferenza

La tortura viene ancora praticata nel mondo e sono migliaia gli uomini che continuano ad esercitarla. Secondo stime di Amnesty International negli ultimi tre anni, in oltre 150 Paesi le Forze di polizia locali hanno commesso torture e maltrattamenti e, in in più di 80 casi, tali pratiche hanno provocato decessi. In 50 Paesi nel mondo vengono torturati minori e non deve sorprendere che la tortura avvenga anche laddove vige la democrazia. Essa è praticata nelle carceri così come nelle abitazioni private e colpisce persone di tutte le estrazioni sociali. Ebbene, dal 1984, da quando cioè la Convenzione delle Nazioni Unite ha stabilito che cos'è la tortura, in Italia si aspetta di introdurre

un emendamento al disegno di legge sulla sicurezza,

Pietro Marcenaro, Andrea Marcucci, Francesca Maria Marinaro, Ignazio Marino, Alberto Maritati, Daniela Mazzuconi, Rita Levi-Montalcini, Claudio Micheloni, Colomba Mongiello, Fabrizio Morri, Magda Negri, Francesco Pardi, Achille Passoni, Stefano Pedica, Carlo Pegorer, Oskar Peterlini, Roberta Pinotti, Nino Randazzo, Francesco Rutelli, Gian Carlo Sangalli, Luciana Sbarbati, Anna Maria Serafini, Achille Serra, Silvio Sircana, Albertina Soliani, Luigi Vimercati, Vincenzo Vita e Luigi Zanda. *(Il senatore

vorrei cercare di dare una spiegazione del lavoro che si sta facendo, poiché si tratta di un inasprimento del carcere duro per i reati di mafia e terrorismo. Tale lavoro ha visto impegnato nel tempo il Gruppo al quale appartengo, con iniziative assunte sin dalla fine degli anni Novanta dall'attuale presidente del Gruppo, senatore Maurizio Gasparri,

ma siamo di fronte ad un fenomeno che è ormai chiaro a tutti, che risulta da atti investigativi e da processi in corso. Vi sono soggetti che, reclusi secondo

abbiamo compiuto non serve solo a punire il singolo soggetto, ma deve dare la certezza che dalle carceri non si comanda perché nelle carceri comanda lo Stato e chi è stato condannato, se vuole evitare il carcere duro, ha un altro strumento: non fare più il mafioso e collaborare con lo Stato, dare il proprio contributo a far sì che il cancro terribile delle mafie, che ancora affligge il nostro territorio, venga finalmente sgominato. Questa è la battaglia che proponiamo, il segnale che vogliamo mandare all'esterno. Vedete, colleghi senatori, in queste settimane talvolta le cronache ci hanno consegnato un'immagine distorta di superlatitanti arrestati; mi riferisco, ad esempio, al boss Bernardo Provenzano, che starebbe nella sua celletta del 41-*bis* con la Bibbia in mano quasi in atteggiamento ascetico. Di fronte a queste presentazioni probabilmente qualcuno dimentica che questa è gente che ha sciolto altri uomini nell'acido,

che vide saltare in aria, con metodi da commando terroristico, magistrati come Falcone e Borsellino. E, ancora, si tratta di soggetti che hanno partecipato alle stragi di recente sono stati del 41-*bis* e consegnati alla detenzione ordinaria. Qualcuno di loro, prima che il ministro Alfano firmasse per confermare il regime del 41-*bis*, ha passato il Capodanno insieme agli altri detenuti! Quando i colloqui con i propri congiunti e con i propri avvocati non servono né per difendersi né per abbracciare o baciare un figlio, ma esclusivamente per portare ordini all'esterno, lo Stato ha il dovere di intervenire perché questa usanza cessi. Questo ci stiamo proponendo di fare, con gli errori che fa chi può legiferare, ma con la buona fede e la voglia di liberare il Paese da una ferita terribile per la democrazia. Mi sarei aspettato

come questo bisogna reagire. Probabilmente chi ha compiuto quel delitto cammina libero e tranquillo, perché tanto l'omertà continua a permeare pezzi importanti del territorio. Questo, dunque, è lo sforzo che abbiamo voluto fare, trovando un'intesa la più larga possibile e riconoscendo che, accanto alla nostra iniziativa, c'è stata quella importante dell'opposizione e che si è potuto lavorare senza pregiudiziali rispetto al raggiungimento di un obiettivo che diventa oggi una vittoria del nostro Parlamento, una vittoria dello Stato contro la criminalità organizzata.

una vittoria perché ci consente di dare al Paese uno strumento migliore per tenere le persone al loro posto, non per tenerle isolate

IlGoverno, che è certamente sensibile alla materia, si permette di ricordare che nel nostro ordinamento non mancano le norme incriminatrici di comportamenti

è anche - mi sembra, però, quasi offensivo ricordarlo in quest'Aula - un'aggravante derivante dall'avere questa posizione. Vi è certamente una convenzione delle Nazioni Unite, ma si deve verificare se e fino a che punto

fa seguito ad una tradizione di impegno del Partito radicale sulle tematiche della giustizia anche in Sicilia: nel passato, quando si sono trovati a scegliere tra l'esigenza di rafforzare l'azione dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata mafiosa

Vorrei ricordare però ai colleghi che il fenomeno mafioso in Sicilia è tutt'altro che sconfitto. Ancora in queste ultime settimane, nonostante i segnali positivi ed importanti che si registrano (vorrei ricordare, tra tutti, la posizione coraggiosa assunta da molti imprenditori siciliani e segnatamente da quelli aderenti alla Confindustria siciliana in una battaglia di prima linea contro il pizzo e le estorsioni), sentiamo che il rischio

Troppe volte abbiamo dato segnali in senso contrario: da un canto leggi ed interventi legislativi che andavano in quella direzione, dall'altro comportamenti di fatto

Tutt'altro, quindi, che una situazione di isolamento totale o addirittura di tortura, come qualcuno vorrebbe far credere. Noi vogliamo, allora, che la normativa che è stata varata dalle Commissioni sia accolta e che sia respinto l'emendamento Chiediamo, anzi, che vi sia un'azione efficace nell'interpretazione quotidiana che consenta di evitare quello che oggi è un fenomeno assolutamente inaccettabile. Per queste ragioni, ricordando anche qui l'insegnamento molto forte che Giovanni Falcone consegnò a chi ebbe la ventura di conoscerlo e di stargli vicino, cioè che

Grazie,

accogliere l'invito formulato dal Governo a ritirare i nostri emendamenti. Lo facciamo per due ragioni fondamentali: in primo luogo, perché intendiamo, con il ritiro degli emendamenti e il voto favorevole sul testo così come licenziato dalle Commissioni, sottolineare l'unità Grazie,

in comune; mi riferisco soprattutto al traffico degli immigranti e all'immigrazione clandestina. Segnalare la necessità di avere una centrale unica, in capo alla Procura nazionale, che si occupi anche della materia della prevenzione, della conoscenza e del contrasto al terrorismo è il senso della

Presidente, colleghi, a me piacerebbe vivere in un Paese senza 41-*bis*, senza 416-*bis,* perché questo significherebbe vivere in un Paese senza mafia, senza organizzazioni criminali radicate nel territorio, con forti capacità militari.

era ed è, purtroppo, ancora pesantemente la realtà del nostro Paese. Nessuna forma di tortura e, per cortesia, non citate Paesi dell'Unione europea che hanno un sistema penitenziario che vede il nostro

Abbiamo pensato ad una norma che, nel solco delle decisioni pronunciate dalla Corte costituzionale, riuscisse a contemperare la possibilità di una detenzione rispettosa della dignità umana con quello che era un imperativo categorico, perché la realtà ci ha parlato di omicidi commissionati dal carcere di organizzazioni criminali che continuavano ad essere dirette in maniera assolutamente esclusiva e totale dal carcere. La realtà ci ha parlato di una caduta verticale di tutto ciò dopo l'introduzione dell'articolo 41-*bis* e dico anche, ai colleghi che parlano

il percorso dei messaggi e tante operazioni delle procure distrettuali antimafia sono state realizzate attraverso questi oggi il 41-*bis* è e non può che essere una norma assolutamente presente nel nostro ordinamento. Le modifiche, che sono state realizzate in maniera assolutamente *bipartisan* con un dibattito costruttivo, mirano anche

si verificheranno sul campo i perfezionamenti introdotti in questa occasione.

dovrebbe anche essere esportata in altri Paesi dell'Unione europea, infettati anch'essi dalle organizzazioni mafiose, ma che continuano a non voler adottare strumenti in grado di recidere i legami tra detenuti e organizzazioni che rimangono all'esterno e a non voler adottare una legislazione antimafia italiana, frutto delle intuizioni di Giovanni Falcone, che è all'avanguardia

È stato detto che si vuole colpire al cuore la mafia. Benissimo: non si può colpire al cuore qualcosa con uno strumento che - dite voi - ha dimostrato la sua inefficacia. Iniziamo con legalizzare le droghe, legalizzare e regolamentare la prostituzione, modificare le nostre leggi relativamente all'immigrazione, di modo da dare un colpo al traffico di esseri umani. Tutto questo va contro la vostra vostra visione- che purtroppo è condivisa anche da molti colleghi del Partito Democratico - di punizionismo e panpenalismo. Ciò che occorre è regolamentare fenomeni enormi per non far diventare le nostre proibizioni qualcosa di criminogeno.

Allora mi dovete spiegare per quale motivo la modifica dell'articolo 41-*bis* prevede che le ore d'aria per un detenuto regime devono passare da quattro a due. Che cosa c'entra? Che cos'è questo se non un andare contro l'articolo 27 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»?

vorrei brevemente argomentare tale mia posizione. Gli sforzi che bisogna compiere per dare certezza alla pena non possono mai travalicare la dignità della persona. Gli sforzi che le Commissioni hanno compiuto per scrivere una norma che contemperasse il diritto di alcuni con il diritto di tutti sono notevoli e apprezzabili, ma certamente sul regime di cui all'articolo 41-*bis* bisognerà molto discutere. Gli sforzi compiuti dai firmatari degli emendamenti in questo senso sono altrettanto apprezzabili ed importanti, ma nessuno né nel caso della formulazione del testo dell'articolo, né nel caso della formulazione del testo degli emendamenti - ha tenuto conto di un dettaglio,

un'attenzione e uno studio specifico, ma in questo momento non c'è dubbio che dobbiamo far prevalere i diritti di tutti prima di far prevalere i diritti di qualcuno. In questo momento, pertanto, pur non volendo esprimermi

Credo che la tortura non sia solo quella fisica e che lo Stato non debba mai avere paura di se stesso. Credo che lo Stato non possa permettere a qualche

come quello sulla tortura. Anch'io sono presentatrice di un disegno di legge sulla tortura; sottoscrivo le dichiarazioni sia della collega Poretti che del collega

e, diciamo, all'80 per cento nelle dichiarazioni che hanno fatto i colleghi radicali Poretti e Perduca. Pertanto, il mio voto è di astensione. [DI

Grazie,

persone come Battisti si registra nel fatto che, dopo la fine dell'emergenza, questo Stato ha trovato nuovamente le condizioni di civiltà. Noi siamo più forti di Battisti e di quelli che la pensano come lui per queste condizioni di civiltà e dobbiamo e possiamo esserlo anche contro la mafia e le criminalità.

Signor Presidente, ho dedicato gran parte della mia vita, anche dal punto di vista professionale, alla lotta e al contrasto al crimine organizzato. Continuerò a farlo fino alla fine dei miei giorni.

Il suo rigore deve essere contemperato rispetto alle esigenze reali. Ferma restando tutta l'impostazione, nella quale mi ritrovo, non posso però condividere la modifica della competenza perché non solo non serve, ma rischia di incidere negativamente sul sistema democratico del giudice naturale. Non possiamo dire - proprio la motivazione del collega Centaro mi ha messo ulteriormente in allarme - che, poiché c'è il pericolo di sentenze diverse e diversificate (ovvero la pluralità e la diversità delle motivazioni), concentriamo tutto sul tribunale di Roma. Questo è un *vulnus* e può costituire un precedente gravissimo. Inoltre, non posso accettare la riduzione dalle quattro

siamo perfettamente d'accordo e abbiamo anche condiviso quasi interamente il testo Grazie,

non ci sarà mai la possibilità da parte del Sud di riprendere una propria vitalità e di dare il proprio contributo alla rinascita economica del nostro Paese se prima non si intraprende una lotta seria, decisiva e determinante nei confronti di tutte le forme di criminalità organizzata. Ben venga quindi tutto ciò che serve alla lotta alla criminalità organizzata. E noi siamo felici felici di votare in questo senso. Per quanto riguarda la tortura, vorrei dire al senatore Mantovano che questo reato, così com'è stato c'era stato un invito da parte delle Nazioni Unite, era stato già preso in considerazione nella scorsa legislatura; il relativo

ma certamente, come ha già detto qualcuno, ciò che non serve dovrebbe comunque essere cancellato. E ciò che non serve è l'abuso dei mezzi di costrizione fatto nel momento in cui si è già rilevato

i Paesi civili hanno introdotto, mi sembra sia una contraddizione veramente grave, che mette in discussione la nobiltà di intenti politici liberali o liberistici che il Popolo della Libertà o il centrodestra stanno contrabbandando nel Paese. Volete uno Stato liberale o volete uno Stato di polizia? Volete uno Stato liberale che garantisca i diritti civili e umani e pene adeguate in linea con una giustizia severa e giusta o volete un inasprimento tanto per far bella la faccia di chi pretende di difendere la giustizia e i cittadini attraverso comportamenti veramente offensivi e lesivi della dignità umana e dei diritti di ciascuno?

Condivido l'ispirazione e le finalità del 41-*bis* e condivido l'opinione espressa poc'anzi dal senatore D'Ambrosio, cioè che il 41-*bis* non abbia nulla a che fare con il tema della tortura.

34, a cominciare dalla previsione del dimezzamento delle ore d'aria. Ritengo, inoltre, inaccettabile il riferimento alla possibilità di riaprire istituti penitenziari speciali nelle piccole isole, a Pianosa come all'Asinara. Per queste ragioni mi asterrò.

Presidente, intervengo per annunciare la mia astensione dal voto perché trovo davvero pittoresco che nel momento in cui nel Paese c'è un grande allarme per la criminalità vi sia un numero così elevato di parlamentari che avvertono l'esigenza di introdurre un reato proprio nei riguardi delle Forze di polizia: il reato di tortura.

Poretti. L'argomento centrale che ci ha portati a proporre l'emendamento soppressivo dell'articolo 34, che non è il sostegno alla criminalità organizzata, che non è una denuncia sull'operato delle forze dell'ordine, ma che è il tentativo di recuperare un minimo di dignità, di civiltà e di speranza nella possibilità che, attraverso lo Stato di diritto, si possa sconfiggere la criminalità e non attraverso la punizione sistematica. Dall'inizio di questa legislatura ci sono state proposte esclusivamente delle misure che vanno nella direzione dell'inasprimento della pena per qualsiasi cosa, in un contesto in cui la certezza del diritto è denunciata quotidianamente dalla Corte di Strasburgo dei diritti umani. Tutto questo, secondo noi, non è il modo con cui si può combattere la criminalità organizzata tant'è vero che dopo 17 anni di 41-*bis* ci è stato detto da più parti che non si è riusciti ad arrivare al cuore della mafia. Concludo ricordando ai compagni del Gruppo del Partito Democratico che nella scorsa legislatura si era tentato di chiudere le due le due carceri minori nelle isole con tutta una serie di motivazioni che andavano dall'economico al civile fino all'ambientalista. Ecco, con questo articolo, voi le farete riaprire. Quindi, il voto è contrario.

grande importanza ai fini del contrasto contro la criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Credo che con questo voto il Parlamento abbia dato un fortissimo segnale al Paese di come il contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata postuli l'esigenza di una convergenza di di tutte le forze politiche o, quantomeno, di una stragrande maggioranza di forze politiche. La Presidenza non può che compiacersi della quasi unanimità di tale voto*.

Se il sottosegretario Mantovano mi chiede di impegnare il Governo a portare a termine il processo di ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura

non capisco allora di cosa stiamo parlando, perché questa materia, come ricordava bene prima il senatore D'Ambrosio, è già stata sviscerata; è già stato approvato approvato all'unanimità dalla maggioranza di allora e dall'opposizione di allora (oggi a parti invertite) esattamente quell'articolo del codice penale che prevede l'introduzione del reato di tortura. Quindi, vorrei chiedere anzitutto lumi al Sottosegretario. Presidente, ripetendo quanto già riferito in precedenza, la posizione del Governo è la seguente. Il Governo ritiene che il protocollo aggiuntivo alla Convenzione ONU sulla tortura trovi già ampia attuazione nell'ordinamento italiano. Non si tratta di una sola norma che reprime fatti qualificabili come tortura, ma di uno spettro di norme che vanno, come prima si ricordava, dalle lesioni personali alle minacce, alle violenze private, per le quali, se commesse dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico, è prevista anche una specifica aggravante. L'ordine del giorno (che non chiedo, evidentemente: invito chi ha formulato questo emendamento, se lo ritiene, a presentarlo in sua vece) va nella direzione di verificare il Governo si impegna attraverso i propri uffici a farlo - se nelle maglie dell'ordinamento c'è qualche sezione che ancora non è coperta dalle norme vigenti in termini di repressione degli abusi dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio.

per garantire che non c'è un'indicazione specifica e che è la tortura che vogliamo estirpare e non semplicemente colpire chi eventualmente sbaglia in un settore.

come un'aggressione alle Forze di polizia ha una concezione aberrante, insultante in primo luogo per gli agenti di pubblica sicurezza ed i Carabinieri che sono fedeli alla Costituzione e alle

Signor Presidente, vorrei intervenire con grande pacatezza per portare i presentatori di questo emendamento ad un ragionamento che sia anche logico e razionale.

In seconda analisi, ritengo che costruire un reato proprio per autori che siano appartenenti alle Forze di polizia, in un momento in cui nel nostro Paese registriamo la commissione di gravissimi reati, sia non solo ingiusto e improprio,

*(PdL)*. Questo emendamento sottintende una grande demagogia, perché si prevede la punizione con delle pene irrisorie anche fatti gravissimi. Oggi l'abuso contro le persone arrestate, quello che voi chiamate tortura, è punito con sanzioni severissime, per reati che vanno dal sequestro di persona, alle lesioni, all'abuso di ufficio: altro che quattro anni! Voi fate demagogia,

Però deve essere chiaro a tutti che il precetto secondo cui è bandita ogni violenza fisica e morale contro le persone arrestate è nella nostra Costituzione e noi onoriamo la Costituzione del nostro Paese, cari colleghi.

credo che sarebbe il caso, poiché stiamo affrontando un tema particolarmente delicato, che implica anche impegni internazionali del nostro Paese, dimostrare

cui singole persone sono state oggetto di condanna per delitti che hanno commesso abusando della loro funzione di pubblico ufficiale. Ciò che non è consentito è trasformare responsabilità individuali in un ragionamento più generale che si traduca in un processo alle Forze di polizia, alle quali però non si rende un buon servizio quando si pensa che qualsiasi tema debba essere affrontato Credo che la formulazione dell'emendamento proposto dai colleghi Poretti ed altri sia sbagliata tecnicamente e nel merito. Credo sia opportuno che tale tema sia affrontato invece facendo una ricognizione preventiva di ciò che l'ordinamento penale già prevede nel nostro Paese per predisporre una norma che sia equilibrata e che persegua il fine per il quale è stata proposta.

presentazione di una proposta *ad hoc*. Qualora i colleghi insistessero nella votazione dell'emendamento, il voto del nostro Gruppo sarà ovviamente di astensione, proprio in considerazione del fatto che il tema è serio e i colleghi hanno fatto bene a porlo. Credo che non sia il caso di alzare il livello del confronto oltre il limite di ciò che il confronto stesso merita solo per rivendicare paternità o maternità che in questo caso ci portano lontano da una discussione sul merito della questione alla quale dovremmo tutti strettamente e con serietà

che, avendo votato il legislatore ed introdotto il delitto di atti di corruzione giudiziaria, si è voluto andare contro i magistrati. Quindi, mettiamo da parte questo argomento.

nell'ambito delle Forze di polizia o fuori, dovessero commettere siffatti delitti. Saranno proprio i poliziotti onesti a procedere contro i poliziotti disonesti. (E spero che ve ne siano sempre di meno nel nostro Paese).

un cono d'ombra presente nel nostro sistema penale, che non prevede il reato di tortura. Nella scorsa legislatura si ritenne

di tornare al testo originario previsto nella Convenzione di New York, che riguardava espressamente il reato di tortura commesso dall'incaricato di pubblico servizio o dal pubblico ufficiale.

Voglio soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sull'ultimo *incipit* della norma proposta: «Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile». Questa è la manifestazione più evidente che la norma è fatta a tutela delle nostre forze dell'ordine e contro coloro che, approfittando della divisa e del ruolo si allontanano dalla Costituzione.

perché dovremmo formulare un ordine del giorno che non mi pare sia emerso in tutto il suo contorno a seguito del dibattito.

«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». È sulla rieducazione del condannato ci siamo concentrati nel proporre questo articolo aggiuntivo che tratta dell'interdizione dai pubblici uffici. Crediamo che la sicurezza richieda politiche di integrazione. I diritti civili e politici sono universali. Fra i diritti politici, in primo luogo vi è il diritto all'elettorato attivo. L'esclusione di coloro che sono in esecuzione penale, a volte anche dopo molti anni dal fine pena, ossia sino a che non interviene la riabilitazione, configura un'ingiustificata preclusione all'esercizio di uno dei diritti fondamentali dell'individuo. L'emendamento 35.0.100 prevede l'eliminazione della privazione del diritto di elettorato attivo dall'elenco delle pene accessorie. La complessiva serie di effetti che consegue alla condanna continua a rispecchiare un'ottica di esclusione dal contesto sociale e democratico e comunque non di aiuto al recupero sociale della persona che, pur avendo sbagliato e scontato la sua pena, si trova privata di importanti diritti quali, ad esempio, quello dell'elettorato attivo. Tale limitazione non può che costituire uno scoglio insormontabile ai fini di un effettivo reinserimento sociale. Per tale motivo, dunque, è auspicabile l'intervento legislativo con l'approvazione di questo emendamento in un campo che da tempo non subisce modifiche migliorative e che invece registrerebbe effetti positivi proprio nell'ottica di quanto previsto dalla terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione. esame, dunque, tende ad eliminare la privazione del diritto di elettorato attivo dal novero delle pene accessorie e, in particolare, dalle limitazioni attualmente riconducibili all'interdizione dai pubblici uffici

di violenza sessuale, che è posto - come preannunciato anche pubblicamente sulla stampa - a carico dello Stato. Noi abbiamo predisposto una serie di subemendamenti

penso sia possibile arrivare al consenso, quanto meno su questa parte che concerne i morti a causa del lavoro.

cosa che credo in queste giornate non debba che vederci tutti assolutamente favorevoli.

Colleghi, la senatrice Adamo ha il diritto di poter esprimere le sue opinioni ed illustrare le sue proposte di modifica in un'Assemblea che sia quanto meno attenta. Chi non è attento è invitato a lasciare l'Aula.

le norme che avevamo proposto con i nostri emendamenti sulla violenza sessuale. Se, per una volta, il Governo ci avesse dato ascolto, oggi staremmo per varare una legge che anche su questi argomenti darebbe immediatamente risposta alle attese della popolazione.

è in modo eclatante riduzione in schiavitù. Peraltro, poiché l'obiettivo del pubblico patrocinio è quello di avere qualcuno che non solo paga, ma prende le difese della vittima e ne tutela il diritto non solo alla giustizia, ma anche a risarcimenti, al reinserimento, all'aiuto ad uscire dalla situazione in cui si è venuta a trovare a causa del colpevole, gli altri nostri subemendamenti cercano di inserire altri reati i quali, sia che si riferiscano alle donne, sia che si riferiscano ai minori, hanno la stessa caratteristica dell'emendamento del relatore, che si riferisce solo ed esclusivamente al reato di violenza sessuale. Vi sono altri reati in cui il pubblico patrocinio per la vittima è garanzia non solo di possibilità economiche, ovviamente, e quindi diritto

legato alle organizzazioni criminali. Si tratta di un fenomeno relativamente al quale forme e misure di prevenzione sono importantissime, quanto anche forme di sostegno soprattutto a chi decide di denunciare. Pertanto, il gratuito patrocinio ci sembra un elemento importante e fondamentale che può servire ad incoraggiare e a sostenere tutte le persone che decidono, eventualmente siano incorse in questo tipo di legami o in questo tipo di

Tante misure come quelle che furono attuate per l'articolo 18 andrebbero fortemente finanziate e riguardano anche i programmi di prevenzione e protezione per chi denuncia gli sfruttatori e i soggetti che fanno uso di questo reato, cioè della tratta degli esseri umani, in particolare praticata sulle donne e sui bambini. Sono forme di prevenzione importantissime perché consentono anche di proteggere le vittime che denunciano e quindi permettono anche di incentivare la collaborazione nei confronti dello Stato. Un'altra incentivazione importante è rappresentata dal gratuito patrocinio. Per questo motivo ci permettiamo di insistere sull'emendamento in esame ritenendolo anche di valore simbolico. Comprendiamo il tema economico, ma non crediamo peraltro peraltro che questo emendamento richieda un apporto molto rilevante di risorse economiche. Ci troveremmo di fronte ad una collaborazione molto forte da parte di questi soggetti e in tal caso forse varrebbe la pena

remote, isolate in qualche parte del mondo e che non ci toccassero minimamente, non siano presenti anche nel nostro territorio, perché connesse ad alcuni fenomeni migratori di cui non abbiamo tempo di sviluppare in questa sede le caratteristiche, sia perché comunque sopravvivenze orribili di pratiche mai completamente sradicate anche nel nostro territorio nazionale e tra cittadini italiani. italiani. Il fenomeno più massicciamente vistoso da questo punto di vista è quello relativo alla tratta degli esseri umani collegato o alla prostituzione minorile e non, o alla produzione pornografica e soprattutto pedopornografica.

da questo giro in questi casi si ritrova in un vero e proprio incubo. Non ci sono distinguo, come in altre situazioni, perché parliamo dell'acquisto e della vendita di esseri umani,

fino ai fenomeni di cui parlavo prima. Quando ci si trova di fronte a questi fenomeni e quando la vittima é stata individuata dalle forze dell'ordine e, a seconda dell'età,

di cui all'articolo 630 del codice penale che disciplina la fattispecie del sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione. La ragione di questo emendamento sta nelle considerazioni che il collega Casson e gli altri hanno presentato per tutti gli altri emendamenti. Nel caso specifico si comprenderà come questo sia un reato fortemente limitativo della libertà della persona; quindi, per questa ragione, ne individueremmo

Basta guardare i dati per rendersi conto che si tratta di un fenomeno che anziché diminuire continua giorno dopo giorno a crescere. Non ultimo, in questi due giorni, si sono verificate altre violenze sessuali. Come già ricordavo la settimana scorsa, in occasione del mio intervento sul fenomeno della violenza contro le donne, secondo il rapporto ISTAT del 2006, erano 6.743.000 le donne dai 16 ai 70 anni ad aver dichiarato di essere rimaste vittime di molestie o violenze fisiche, psichiche o sessuali nel corso della propria vita. Di queste circa un milione ha subito stupri o tentati stupri. Purtroppo, nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate. Ciò che possiamo definire come il sommerso è tuttora elevatissimo. La violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenni, la violenza sessuale di gruppo sono reati aberranti che scuotono le coscienze personali e provocano un senso diffuso di paura e di insicurezza nella cittadinanza. di reati che, se pure da un lato violano la sfera più personale ed intima, dall'altro lato colpiscono in modo indiscriminato l'intera comunità cittadina, provocando sdegno e un sentimento diffuso di ingiustizia. Nel momento in cui un balordo violenta una donna o un bambino, o peggio ancora un gruppo di sciacalli si accanisce su una vittima indifesa violandola o provocandole ferite, che soltanto Dio sa quando potranno essere riemarginate, qualunque pena appare lieve e sproporzionata al reato. Gli ultimi fatti di cronaca confermano quindi che la violenza fisica e sessuale rappresenta ancora oggi una delle forme di violazione dei diritti umani più grave e diffusa nel mondo e nel nostro Paese, che produce effetti devastanti sulla vita di tutti. Spetta quindi a tutti i Governi nazionali adottare misure rigorose per arginare tale fenomeno e per tutelare i diritti degli individui, come chiede anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La gravità del fatto e il rispetto della dignità delle vittime impongono interventi sanzionatori capaci di restituire all'intera società credibilità nella giustizia. Noi politici abbiamo il dovere di dare una risposta concreta; non possiamo e non dobbiamo limitarci esclusivamente a criticare l'operato della magistratura che, seppur nell'esercizio discrezionale, è obbligata al rispetto della legge. Se di fatto la normativa vigente permette di concedere la custodia cautelare agli arresti domiciliari ad un reo confesso di violenza sessuale, che trova come uniche giustificazioni e scusanti quelle di avere agito sotto l'effetto di alcool, droga o quanto altro, noi legislatori non possiamo fare altro che apportare le giuste modifiche anche perché tanti colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, hanno dichiarato che non bisogna concedere la libertà provvisoria o forme di detenzione alternativa nei casi di gravi reati come la violenza sessuale. Inoltre, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha dichiarato ieri che lo stupro è un delitto imperdonabile ed esecrabile e scarcerare gli autori, come deciso dal GIP di Roma e Guidonia, è da considerarsi un errore. Qualche giorno fa gli stessi magistrati hanno ritenuto di prevedere la custodia cautelare agli arresti domiciliari per Davide Franceschini, indagato nella inchiesta sullo stupro, avvenuto nella notte di Capodanno a Roma; hanno dichiarato che quando il legislatore restringerà il potere del giudice questi agirà di conseguenza. nuova formulazione, va in questo senso, onorevoli rappresentanti del Governo, mirando ad escludere la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni e la violenza sessuale di gruppo dalle fattispecie di reati per i quali agli imputati possono essere concesse misure alternative alla detenzione. Inoltre, la nostra proposta prevede che per i reati di violenza sessuale sia sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere,

rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, credo che questa non sia una soluzione, però penso che abbiamo il dovere, una volta tanto,

che si fanno su questi argomenti, bensì intervenendo con la legge in modo che anche la magistratura non possa dire che sono i legislatori a dover intervenire. Noi lo chiediamo con forza.

Si tratta di un emendamento di grandissima attualità che credo possa trovare la condivisione dell'intera Aula del Senato. Con questo emendamento i relatori propongono che i soggetti vittime dei reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni e di violenza sessuale di gruppo possano sempre chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche qualora i propri redditi superino le soglie previste dalla legislazione vigente, in considerazione della particolare efferatezza delle fattispecie criminose in oggetto e della evidente influenza nel tessuto sociale delle relative condotte lesive a cui ogni giorno la carta stampata e la televisioni Questo nostro emendamento viene riformulato dai relatori (e, conseguentemente, tutti i subemendamenti dovranno essere ricollocati sulla nuova riformulazione)

L'aggiunta che proponiamo in un emendamento più asciutto rispetto a quello precedente è la seguente: «2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

sosterrà questa iniziativa, che è un atto di grande civiltà e di vicinanza soprattutto nei confronti di quelle persone che, tragicamente, muoiono

che obblighi ciascuno di noi ad una riflessione nella doppia veste di cittadini e di legislatori, ma forse ancor di più di genitori, di fratelli, di sorelle, di figli di donne che possono trovarsi nella drammatica situazione di subire una violenza spesso inaudita. A questo fenomeno assistiamo, purtroppo inermi, da troppo tempo ma è innegabile che l'allarme sociale che si sta determinando nel Paese riguardo a questo tipo di reati ci obbliga ad una riflessione tempestiva. Non voglio entrare necessariamente nell'ambito difficile, complesso e sottile del diritto perché le discussioni sarebbero lunghe. Il presidente Berselli prima ci ha intrattenuto in modo assai interessante su alcune sue considerazioni. Chiedo ai colleghi per un momento di mettersi una mano sulla coscienza e di rispondere da legislatori, cittadini, genitori, figli, fratelli, sorelle a questa emergenza che si va determinando nel Paese per due motivi fondamentali, a mio modesto avviso: una cattiva interpretazione del ruolo della magistratura in queste vicende che mette in luce, insieme ad altri aspetti, il fallimento del nostro sistema giudiziario, perché là sta il vero e grande problema. Ormai il tema della giustizia è una vera e propria emergenza nel Paese, sia che esso riguardi la giustizia civile come quella penale e tutti lo vivono sulla propria pelle, dai cittadini innanzitutto alle imprese alle istituzioni. Quanti enti locali sono bloccati e rallentati nei processi civili ed amministrativi? Quante imprese subiscono danni da una giustizia civile che non funziona e, ahimè, quanti cittadini pagano sulla propria pelle una giustizia che ormai in questo Paese è diventata un sepolcro imbiancato? Il secondo aspetto che a me interessa mettere in evidenza, forse ancora di più nell'ambito di questa discussione, è che è che c'è dietro questo fenomeno una preoccupante deriva culturale, che deve farci interrogare sui vuoti che abbiamo contribuito a determinare nel sistema dei valori, nella trasmissione dei nostri valori alle giovani generazioni, a quelli che poi improvvisamente conosciamo come dei ragazzi normali ed improvvisamente scopriamo essere un branco o dare vita ad un branco. o dare vita ad un branco. C'è un grande lavoro che tutti noi dobbiamo poter fare a partire da qui, senza aspettare che lo facciano altri, senza aspettare che altri cerchino di difendere come possono ciò che hanno e soprattutto facendo in modo che non si ingeneri nella coscienza civile di questo Paese la certezza che lo Stato non dà certezza, e non solo della pena, ma nemmeno dell'intervento, e la certezza ancor più pericolosa per tutti noi che ci dobbiamo arrangiare e farci giustizia da soli. Le reazioni che in questi giorni abbiamo visto verificarsi in alcune situazioni (Guidonia per esempio, ma ve ne sono molte altre che non cito e che non è così importante citare) segnalano però che i cittadini sono stanchi di sopportare mille vessazioni, di non veder riconosciuti i propri fondamentali diritti - e la sicurezza è un fondamentale diritto dei cittadini che si uniscono in una società, in uno Stato, in una comunità e sono ormai determinati a farsi giustizia da soli. Se non vogliamo da domani dover affrontare anche altri drammatici problemi, abbiamo l'obbligo, senza necessariamente rincorrere l'emotività suscitata dai *mass media*, *mass media*, di sapere, di conoscere che questo fenomeno sta determinando un allarme vero, culturale e sociale, nel nostro Paese. Se noi siamo legislatori responsabili, abbiamo il dovere di anticipare per una volta e non di rincorrere sempre: l'inasprimento delle pene rispetto a questo tipo di violenze ormai non è più rinviabile. Così come non è più rinviabile una discussione approfondita, non solo da parte nostra ma di tutti i protagonisti di questa società, sempre più malata e che necessita di un intervento culturale prima ancora che normativo, rispetto al dialogo con i genitori e con la scuola, con gli attori protagonisti che sono alla base della vicenda umana della nostra società. vicenda umana della nostra società. Se ci dimentichiamo questo allora le nostre leggi, le nostre norme, anche se buonissime, resteranno scritte sulla carta e basta. Faremo ottime leggi per la carta. La realtà non sta però nella carta, sta fuori di qui: e fuori di qui, questo Paese non vive più bene. Non vivono più bene le donne di questo Paese, costrette a fare i conti con un problema di sicurezza che condiziona pesantemente la loro vita, e ancora troppo spesso costrette a fare i conti con un'arretratezza culturale che ci ha portato finora a sottovalutare in modo colpevole (voglio dire criminale) criminale) tale dramma, che pensiamo sempre appartenga ad altri. Ormai i dati statistici ci dimostrano però che gli altri cominciamo ad essere noi e che in ogni nostra famiglia può verificarsi un evento così drammatico, drammatico, dentro e fuori le mura domestiche. L'appello alla coscienza di tutti noi forse servirà oggi a farci votare non una norma in più, non solo un inasprimento, ma una svolta culturale in tema di rispetto delle donne, che solo una stigmatizzazione di quel segnale che ci viene richiesto di forte punizione di chi mette in discussione la sacralità del corpo e dell'animo femminile.

è oggi Presidente di turno

forse perché non c'è la consapevolezza di una crisi. Ho chiesto anche al mio Capogruppo che la questione venga portata alla Conferenza dei Capigruppo, perché era stata già calendarizzata. Più di una volta, abbiamo riproposto che venisse messa in discussione e ci auguriamo

Ci sono industrie che stanno chiudendo, lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro, famiglie indebitate.

In questi giorni, in particolare ieri e questa mattina, il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi, ha ritenuto di dover interferire in maniera gravissima sullo svolgimento delle elezioni regionali in Sardegna. Lo ha fatto assumendosi la gravissima responsabilità di proferire parole a dir poco ingiuriose nei confronti del candidato del centrosinistra, l'onorevole Renato Soru. Basta leggere i giornali di oggi, ma ciò sarà possibile anche guardando i giornali di domani, o ancora meglio guardando le registrazioni di una trasmissione andata in onda ieri su "Rete4" e quelle di un'altra che andrà in onda oggi su "Canale5", per rendersi conto di quale tasso di impudenza, di arroganza di inadeguatezza istituzionale il Presidente del Consiglio abbia saputo esprimere, permettendosi di valutare, sia dal punto di vista politico che da quello etico e morale, il candidato del centrosinistra. Mi rendo conto che apparentemente, signora Presidente, in una società in cui conta la comunicazione - e io sto parlando con

ha potuto scorrazzare senza alcun rispetto della *par condicio*. Tuttavia, per essere fedele e leale al significato di questo intervento, la prego, signora Presidente, di intervenire sul Ministro dell'interno per chiedergli di considerare la necessità di sviluppare le opportune iniziative per eliminare, o quantomeno contenere, i pericoli di tipo politico ed elettorale che la protervia e l'arroganza del Presidente del Consiglio stanno determinando. Ciò al fine di favorire un normale, regolare, serio svolgimento delle consultazioni elettorali, che anche in Sardegna debbono potersi svolgere come altrove. *(Applausi dei